non con l'inevitabile metro delle aspettative o, nel caso di questo Governo, con quello un po' taroccato della retorica, ma con il metro della realtà dei fatti. Con questa "prova del nove", i programmi, i dati previsionali e gli obiettivi dichiarati sono sottoposti a verifica per appurarne il grado di realizzazione e, quindi, l'attendibilità di chi ha sostenuto quei programmi e quelle previsioni ed ha individuato quegli obiettivi. Così, per l'Esecutivo, e purtroppo per l'intero Paese, questo autunno è uno dei primi momenti delle grandi verità. Dopo il dato estivo di Banca d'Italia, che ha ufficializzato il nuovo *record* del debito pubblico, che ha toccato quota 2.241 miliardi, dovendo arrendersi all'evidenza, solo qualche giorno fa il Governo ha dovuto rivedere al ribasso le previsioni del quadro macroeconomico previsto nel DEF di primavera. Una modifica tutt'altro che marginale, nonostante le rassicurazioni di ieri del ministro Padoan, che costringerà il Governo ad una manovra spericolata, sottoponendo quindi ad ulteriori sacrifici il Paese, per rispettare gli impegni europei e continuare a sostenere che i conti pubblici sono a posto e che la nostra economia si è incamminata sul sentiero della ripresa.

delle scelte di bilancio al risanamento della finanza pubblica. E questo non per un pregiudiziale atteggiamento di ostilità o per una sterile voglia di opposizione a tutti i costi, che certamente non appartiene al Gruppo dei Conservatori e Riformisti. Il giudizio negativo che esprimiamo - e non siamo solo noi a farlo - si basa sulle risultanze della gestione dei conti statali, che risultano certamente insufficienti rispetto a quelle necessarie a raggiungere gli obiettivi prefissati. Basterebbe vedere le poste che sinteticamente esprimono l'andamento di tali conti, i risultati differenziali, quelli più sensibili per l'Europa: un *deficit* a meno 2,6 per cento, un risparmio pubblico tornato in negativo dopo diversi anni ed un avanzo primario che rimane in territorio positivo, ma di poco, indietreggiando pericolosamente dai circa 30 miliardi del 2014 ai poco più di 2 miliardi E sull'avanzo primario si sono spese in quest'Assemblea milioni di parole negli anni passati. Ma la nostra contrarietà al documento governativo non si ferma al dato in sé. Una lettura più approfondita delle risultanze contabili, basata sulla composizione delle poste attive e passive, dimostra come i risultati della gestione, ancora una volta, siano ben lontani da quelli che il Governo aveva prospettato. Mi limito a considerare solo alcune delle numerose criticità. Per quanto riguarda le entrate, è certamente interessante il dato relativo all'ammontare delle risorse complessivamente affluite all'erario. Il Governo enfaticamente evidenzia come la gestione delle entrate dello Stato sia stata caratterizzata, in positivo, da un gettito complessivo che si attesta a circa 570 miliardi, ovvero quasi 20 miliardi in più di quanto previsto. Ma credo che non dovremmo essere così contenti. Infatti, andando a vedere meglio il dato delle entrate finali si vede come a quel segno "più" concorrano significativamente le entrate tributarie, in aumento di circa il 2 per cento rispetto al 2014, e in particolare IRPEF e IVA,

nel 2015 i complessivi 7,7 miliardi, con una flessione rispetto all'anno precedente del 3,9 per cento, sono stati attinti sempre dai soliti noti, ovvero da chi è già conosciuto e che con grande difficoltà sopravvive non solo alla crisi, ma alla voracità di questo Stato. Questa situazione complessiva sta a significare che l'incremento del gettito erariale non deriva dai marginali incrementi del PIL, dai faticosi "zerovirgola" con cui ci siamo purtroppo abituati a misurare l'incremento della nuova ricchezza. Il gettito per l'erario per l'erario cresce grazie all'ulteriore ed ennesimo sacrificio imposto ai cittadini, alle imprese ed alle parte produttiva del Paese: peraltro sempre i soliti noti, dato che non è chiaro quando e come sia possibile un allargamento della base imponibile ad ambiti personali e settoriali, ad oggi ancora sconosciuti o solo parzialmente conosciuti al fisco. Quindi si rassegnino gli artigiani, le piccole imprese e il commercio di questo Paese; saranno solo loro, insieme ai professionisti e al lavoro autonomo, gli unici ad essere davvero tassati, quando non tartassati. Una situazione che può essere riassunta emblematicamente anche dal settore immobiliare; una cartina di tornasole della situazione economica complessiva. A partire dal Governo Monti, i Governi hanno inopinatamente sposato l'idea, sostenuta fortemente da molti esponenti di questo Governo e anche in sede europea,

Tutto ciò a fronte di persistenti fenomeni di evasione e di erosione della base imponibile che, secondo alcune stime, «evapora» per un importo dal 15 per cento al 30 per cento circa. Sul fronte delle spese, però, la situazione è più chiara e, soprattutto, più preoccupante. L'aumento della spesa è indiscutibile, anche volendo considerarla al netto delle regolazioni contabili. La sua flebile contrazione rispetto al «previsto» lascia il campo al tangibile e concreto aumento rispetto al 2014 - la spesa aumenta persino rispetto al 2014 - nei suoi diversi aggregati «di competenza»: la spesa complessiva cresce del 3,5 ancora di più quella corrente al netto della spesa per interessi che raggiunge il più 11,5 per cento. La spesa aumenta dell'11 sono solo le uniche spese che avrebbero un senso se davvero si volesse rilanciare il Paese verso la ripresa; quella spesa in conto capitale avrebbe un senso e un grande significato per un Paese che volesse tornare a crescere. Invece quella è diminuita del 42 la metà degli investimenti previsti sono stati ridotti, il che vuole dire che senza investimenti è quasi certo che non ci sarà alcuna ripresa. Presidente, concludo questo mio intervento in discussione generale, richiamando l'attenzione di quest'Assemblea, ma soprattutto del Governo, a svolgere un'analisi seria e a non continuare a raccontare favole su conti dello Stato che non sono quelli che racconta il presidente del consiglio Matteo Renzi; sono conti molto più amari, e spero nella nostra dichiarazione di voto di riuscire a portare ulteriori elementi per

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, essendo ormai passati trentuno mesi dall'insediamento del Governo Renzi, la lettura del Rendiconto per il 2015 e dell'Assestamento per il 2016 vada fatta unitamente all'esame dei documenti di contabilità pubblica sinora prodotti. Ricordo che stiamo valutando dei dati sui conti pubblici appena revisionati dall'ISTAT e dalla Nota di aggiornamento al DEF appena pubblicata. Questi dati ci testimoniano quanto è stato realizzato, basandosi sui numeri e quindi sui dati oggettivi, da cui non si può prescindere per arrivare a un giudizio sulla politica economica di Le tre manovre economiche, decreto-legge n. 66 dell'aprile 2014, legge di stabilità del dicembre 2014, legge di stabilità del dicembre 2015 sono state realizzate in *deficit*. Questo ha comportato l'emissione di nuovi titoli pubblici e fatto crescere lo *stock* del debito pubblico, giunto al suo *record* storico di 2.252 miliardi di euro a luglio 2016. Ricordo che era 2.067 miliardi nel febbraio 2014, quindi 185 miliardi in meno da quando il *premier* Renzi si è insediato. A presidio delle coperture finanziarie delle manovre sono state, via via, introdotte clausole di salvaguardia sulle imposte e sulle accise. Quelle attualmente pendenti valgono complessivi 56 miliardi (15 miliardi nel 2017, 20,5 miliardi Nelle manovre sono state introdotte alcune misure *una tantum*: nel 2014, 1.800 milioni di euro di imposte sulle partecipazioni delle banche nella Banca d'Italia; varie imposte sostitutive; nel 2016, oltre 4.000 milioni derivanti principalmente dalla tassazione dei capitali italiani detenuti all'estero. La riduzione delle tasse vale circa 47,8 miliardi. Ma al contempo l'aumento delle tasse, anche

Quindi non comprendo come si possa parlare - come peraltro riportato dai giornali - di «un impegno di riduzione delle tasse che non ha paragoni nella storia del Paese», come sentiamo ripetere quasi ossessivamente dal Governo. La celebrata riduzione della spesa pubblica, pari in totale a circa 42 miliardi, è stata per metà a carico degli enti territoriali (21 miliardi a carico di Regioni, Province e Comuni), e per l'altra metà è stata a carico dello Stato centrale. Ma è evidente come il valore della riduzione di spesa dei territori abbia registrato una contestuale diminuzione dei servizi resi nei confronti dei cittadini a livello locale. Anche la riduzione della spesa è stata ampiamente superata

Se ne deduce un aumento complessivo della spesa per 35 miliardi di euro riferibili alle misure adottate dal Governo Renzi. Della dinamica della spesa corrente sono testimoni i due disegni di legge al nostro esame: la spesa sale di complessivi 43 miliardi tra il 2013 e il 2016. Si tratta, quindi, di manovre fatte a carico delle generazioni future attraverso un aumento dell'emissione dei titoli di Stato e creando, come ho detto poco fa, il *record* storico del debito pubblico.

ma è salito meno rispetto ad altri Paesi europei, registrando in Italia una crescita dello 0,7 per cento nel 2015. Il PIL è infatti passato dai 1.620 miliardi del 2014, ai 1.642 del 2015. questo significa che le manovre economiche renziane hanno avuto in realtà un effetto depressivo sul PIL, che si può calcolare in almeno 18 miliardi tra il 2014 e il 2016, se il PIL arriverà a 1.672 miliardi, come è nelle previsioni.

Quindi in tre anni il Governo Renzi ha ricevuto un regalo cumulato quantificabile in quasi 24 miliardi di euro. L'azione del Governo ha trasformato questo regalo in una crescita della spesa, in particolare di quella corrente. L'azione della BCE, purtroppo, ha favorito quello che non doveva succedere, un allentamento delle politiche di rigore sui conti pubblici italiani. E nel momento in cui l'aiuto della Banca centrale dovesse finire, gli oneri sul debito pubblico potrebbero diventare veramente insostenibili per il nostro Paese. Gli interessi andranno calcolati su un debito che è cresciuto di 345 miliardi dal 2011, l'anno della speculazione dei mercati sul nostro debito pubblico e dello *spread* con i *bund* tedeschi oltre i 500 punti base; l'anno in cui il debito ammontava a 1.907 miliardi.

La mancanza di fiducia nell'azione di questo Governo si è anche palesata attraverso il *gap* tra investimenti esteri in Italia e investimenti italiani all'estero: un aumento di circa 150 miliardi degli investimenti italiani all'estero e una diminuzione di 28 miliardi di quelli esteri in Italia nei tre anni di Governo Renzi. Il flusso di liquidità proveniente dalla Banca centrale europea arriva in Italia e viene investito all'estero, segno evidente di questa sfiducia. Infine, il mancato impegno sulla revisione della spesa ci rende ancora di più la fotografia di questo Governo dalle politiche allegre. Tutti i numeri stanno a dimostrare che siamo di fronte non a un Governo illuminato, ma a un Esecutivo che adotta politiche di *bonus*, a caccia del consenso di brevissimo periodo.

Capisco che le opposizioni calchino la mano sulle leggere differenze, ma, complessivamente, quanto previsto dal DEF e dalla legge di stabilità è sicuramente confermato dall'assestamento. anche il DEF presentato in questi giorni contiene alcuni aspetti che lo confermano. Vi sono misure che ritengo estremamente importanti, la recente legge delega sulla lotta alla povertà, che ha introdotto il reddito di inclusione: una misura di sostegno economico accompagnata da servizi personalizzati con l'inclusione sociale e lavorativa.

Veniamo ora ad alcune considerazioni metodologiche, perché gli interventi che mi hanno preceduto non hanno forse fatto chiarezza. Il disegno di legge di assestamento in esame ha il suo principale riferimento normativo nell'articolo 33 della legge di contabilità e finanza pubblica. La norma dispone che, entro il mese di giugno di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenti al Parlamento un disegno di legge per l'assestamento, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto nell'esercizio concluso il 31 dicembre dell'anno Quindi, ciò che facciamo è mettere in raccordo fra loro strumenti di contabilità diversa. La funzione del disegno di legge di assestamento costituisce lo strumento di aggiornamento a metà anno degli stanziamenti di bilancio determinati in applicazione dei criteri della competenza e della cassa,

In particolare, il disegno di legge di assestamento si connette funzionalmente con il Rendiconto di bilancio relativo all'esercizio precedente e, infatti, l'entità dei residui attivi e passivi sussistenti all'inizio dell'esercizio finanziario, che al momento dell'elaborazione e approvazione dei bilanci di previsione è stimabile

luogo, la relazione illustrativa esplicita che il disegno di legge di assestamento tiene conto degli effetti finanziari derivanti da tutta la riforma delle banche di credito cooperativo,

altro punto importante. Il saldo netto da finanziare presenta una variazione di segno negativo dovuta a un peggioramento di 1.337 milioni di euro per atti amministrativi, ma anche un miglioramento di 243 milioni di euro associato proprio alle proposte dell'Assestamento stesso. Ne risulta che, a fronte della previsione iniziale della legge di bilancio, il saldo netto da finanziare nelle previsioni assestate si attesta su un valore di meno 35.000 di euro, con un peggioramento del 3,2 per cento. Questo è comunque un valore poco al di sotto del limite massimo stabilito dalla legge di stabilità per il 2016, fissato in 35.400 milioni di euro. di euro. Vorrei poi sottolineare che nella proposta di assestamento si determina un miglioramento del saldo netto da finanziare, in modo particolare ascrivibile a una importante riduzione della spesa per interessi Questo è estremamente positivo e sconta l'aggiornamento del profilo dei tassi d'interesse sui titoli pubblici, con conseguente riduzione della spesa per interessi di oltre 3,4 miliardi e riduzione degli interessi passivi Altro aspetto che vorrei sottolineare è che la maggiore spesa è legata anche all'incremento dei trasferimenti alle Regioni, principalmente all'adeguamento delle spettanze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in relazione all'andamento delle entrate erariali. proposito la relazione sottolinea come queste variazioni siano positive per gli enti locali. le riduzioni apportate alle entrate tributarie con il provvedimento di assestamento, si tratta di 2.129 milioni per le imposte dirette e di 1.381 milioni per quelle indirette. A questo proposito vorrei solo sottolineare, in particolare, che abbiamo variazioni di rilievo per l'IRES (375 milioni), le imposte sostitutive sui redditi, nonché su interessi e altri redditi da capitale per 2,2 miliardi, mentre abbiamo delle diminuzioni sull'imposta di bollo e l'accisa sul gas naturale. Si segnalano altresì variazioni in aumento per le imposte sostitutive dell'IRPEF e delle relative addizionali e i versamenti derivanti dall'adesione alla procedura di collaborazione volontaria. Con riferimento alle entrate extratributarie, la variazione in aumento proposta con il provvedimento deriva principalmente dalla partecipazione agli utili di gestione della Banca d'Italia e ai dividendi dovuti alle società partecipate, nonché ai proventi dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche a seguito L'incremento delle spese correnti è dovuto - come dicevo prima - al trasferimento alle Regioni di 3.900 milioni. In particolare, abbiamo un incremento di 4 miliardi di euro di trasferimenti agli enti locali derivati dalla maggiore spesa regionale per oltre 2 miliardi e dall'adeguamento contabile dei fondi per 1,7 miliardi a copertura del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. fatte alcune osservazioni sulle spese in conto capitale, vorrei sottolineare che la proposta di assestamento determina una lieve riduzione di 74 milioni di euro che - devo dire

assegnare al Comune di Roma per il piano di rientro finanziario), con i maggiori contributi agli investimenti delle imprese (1,1 miliardi, di cui un miliardo riferibile a pagamenti residui da erogare a favore delle Ferrovie dello Stato); le acquisizioni delle attività finanziarie il cui aumento delle dotazioni è riferito, per oltre 600 milioni, alle somme necessarie al pagamento dei residui passivi per assicurare agli enti locali la liquidità necessaria per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili.

manovre. Il miglior programmatore dovrebbe avere una sfera di cristallo. Giustamente si prevede un assestamento a metà anno ed è chiaro che il Governo - e con esso la sua maggioranza - crede maggiormente alle previsioni,

scelte di politica economica e fiscale che dovremo compiere a partire dalla discussione e dalle votazioni sulla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza,

riguardo, la mia replica odierna contiene semplicemente un rinvio a ciò che potremmo osservare, dai nostri diversi punti di vista, in sede di discussione sulla Nota di aggiornamento

Il primo ordine di questioni, sollevato da numerosi interventi, riguarda ancora una volta i presunti insoddisfacenti risultati ottenuti attraverso l'operazione che chiamiamo "revisione della spesa". Si è cioè sostenuto che i dati assoluti relativi alla spesa pubblica dimostrerebbero che le operazioni di revisione della spesa non hanno avuto efficacia. Credo che questa valutazione sia il frutto di una vera e propria operazione arbitraria, dal punto di vista logico, di una vera e propria operazione arbitraria, dal punto di vista logico, e anche curiosa sotto il profilo politico, perché una parte di coloro che sostengono questa tesi, secondo cui sulla revisione della spesa, nel corso di tutti questi anni, non abbiamo ottenuto risultati, è stata protagonista di esperienze importanti e durature di Governo, durante le quali sono stati ottenuti risultati positivi nell'operazione di riduzione e revisione della spesa.

ordini di intervento particolarmente incisivi sulla cui qualità, naturalmente, la mia opinione è molto articolata. In termini quantitativi, il primo grande intervento sulla cosiddetta revisione della spesa fu rappresentato dal decreto Tremonti, avvenuto subito dopo la formazione del Governo Berlusconi, dopo le elezioni. Si trattò di un intervento che aveva una portata quantitativa in termini di riduzione della spesa, molto forte e che venne significativamente corretto poi nel corso del lavoro parlamentare successivo, durante il Governo Berlusconi non ho difficoltà a dirlo, anzi sono contento di poterlo dire - anche accogliendo, proprio in questa Assemblea, proposte emendative avanzate dall'allora opposizione, che risultarono incisive per modificare quell'approccio; un approccio che - com'è noto ottenne molti risultati, ma che fu fondato sul metodo del taglio lineare: metodo discutibile e discusso, ha però ottenuto importanti risultati quantitativi. Oggi la spesa pubblica italiana sarebbe decisamente superiore in termini se il decreto Tremonti non fosse stato approvato. Quale sia la ragione per cui quelli che l'hanno pensato e votato adesso neghino questo dato di fatto, a me sfugge, ma in ogni caso così è. Il secondo intervento molto incisivo, soprattutto per una ragione, fu il decreto-legge del Governo Monti, immediatamente successivo alla formazione di quel Governo,

i risultati di quella operazione sono tuttora molto incisivi nei conti pubblici della Nazione, malgrado le diverse operazioni di cosiddetta salvaguardia degli esodati abbiano portato a utilizzare 11 miliardi di quei risparmi, che ammontano però, nel tempo, a diverse decine di miliardi,

può aver mantenuto la stessa opinione, ma è difficile negare che dal punto di vista quantitativo quel provvedimento abbia ottenuto risultati importanti. Terzo e ultimo grande filone di intervento, su cui si sono applicati i Governi nel corso degli ultimi dieci anni, concerne le misure di contenimento tramite razionalizzazione delle spese per acquisto di beni e servizi, che sono state affidate alle cure di diversi commissari che su questo punto hanno ottenuto risultati incisivi, soprattutto grazie all'azione di una struttura pubblica creata a questo scopo - come sapete, è la Consip - che ha fatto sì che gli acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione potessero svilupparsi in maniera decisamente più efficace. gran parte di questi risparmi, che sono stati quantitativamente molto grandi, sia stata impiegata per operazioni di finanziamento di riduzione della pressione fiscale o di nuova spesa - per esempio per fare fronte alle conseguenze della grave recessione nella quale

utilizzato i proventi derivanti dall'operazione di revisione della spesa, ma secondo me è irragionevole - non è fondato sui fatti - sostenere che l'operazione di revisione della spesa non è risultata efficace. Qui semmai - e termino su questo punto

nuova legge di contabilità e l'attuazione della riforma della pubblica amministrazione, per cui sono stati largamente emanati decreti legislativi. La combinazione di queste due riforme strutturali (non solo la riforma della

la politica italiana riuscirà finalmente a fare ciò che non ha mai fatto? Riuscirà a usare per la riduzione e la revisione della spesa anche la valutazione in termini di obiettivi dell'azione amministrativa e del mutamento dei comportamenti, oltre che l'innovazione legislativa? Su questo punto, per ora, non ci siamo, e mi riferisco anche all'attività del sottoscritto e del mio Ministero. Ma la nuova legge di contabilità crea le premesse perché, a partire dal marzo prossimo, su questo punto si sviluppi un'azione finalmente nuova. Il secondo ordine di questioni che voglio molto rapidamente affrontare, avendo riguardato gli interventi riferiti al Rendiconto e all'Assestamento, è il giudizio sulle dimensioni della pressione fiscale in Italia. Si è detto, che i che i numeri assoluti delle entrate dimostrerebbero che il Governo racconta favole quando dice di avere ridotto la pressione fiscale, e sono stati citati i numeri.

risorse derivanti da azioni che fanno acquisire a quelle entrate nuove carattere strutturale - come per esempio dall'azione di contrasto all'evasione - riesco a ottenere un valore x, che non è limitato a un anno, ma si ripete per tutti gli anni. Se, attraverso quelle risorse, faccio un intervento di abolizione dalla base imponibile dell'IRAP della componente "costo del lavoro", non cambio la pressione fiscale totale, perché entrate sono quelle che derivano dal contrasto efficace all'evasione e entrate sono quelle a cui rinuncio quando elimino, dalla base imponibile dell'IRAP, la componente "costo del lavoro". Ma se non guardo all'interno di quel numero relativo alla pressione fiscale vedendo che ho fatto questa operazione, non riesco ad apprezzare un punto fondamentale. L'effetto sul prodotto delle due forme di entrata (sempre 100 di entrata) è molto diverso. Il moltiplicatore positivo della riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sull'impresa è molto elevato (non c'è bisogno di essere un grande economista per capirlo) rispetto ad una entrata che si limita a contrastare l'evasione fiscale che, probabilmente, è un fenomeno che il prodotto, non solo non lo fa aumentare, ma molto probabilmente, tendenzialmente, nel lunghissimo periodo lo fa addirittura diminuire.

quelle risorse che, attraverso entrate aggiuntive, sostituiscono entrate che oggi ci sono e che sono estremamente penalizzanti per le prospettive di sviluppo del Paese. Per esempio, tutto ciò che deriva da pressione fiscale sui produttori, cioè sul lavoro e sulla impresa, certamente ha un effetto depressivo della crescita molto più elevato di quello delle imposte che agiscono su altre base imponibili e, in particolare, molto più elevato delle operazioni di entrata che si realizzano attraverso il contrasto di fenomeni di elusione e e di evasione. forse non è neanche metà dell'opera, perché l'opera sarà conseguita quando sostanzialmente, a parità di livello di pressione fiscale, la pressione fiscale sul lavoro e sull'impresa sarà scesa in Italia alle dimensioni che ha, più o meno, in Germania, mentre avremo realizzato operazioni che sostituiscono queste entrate con altre, la cui presenza ha un impatto negativo sul prodotto, oppure un impatto neutro.

per porre questioni relative al sistema bancario. Io non parlo di singole banche, ma voglio semplicemente ricordare che, per quanto riguarda il rapporto tra bilancio pubblico e sistema bancario, il paese Italia è di gran lunga quello che si

degli effetti ci sarebbero se ciò accadesse, ma sarebbero inferiori a quelli che si determinano in quei Paesi nei quali il bilancio pubblico ha già un'enorme esposizione verso il sistema bancario. Detto questo, noi consideriamo che il complesso di misure adottate nel corso di quest'anno e mezzo, di cui alcune riforme strutturali (riforma delle banche popolari, riforma delle banche di credito cooperativo,

riteniamo di aver fatto pienamente, a questo proposito, la nostra parte.

abbiamo presentato l'ordine del giorno G100 per riprendere un discorso che si era interrotto lo scorso luglio con la legge europea. Sono emerse delle criticità

intervengo per un rapida dichiarazione di voto sugli obiettivi ambiziosi e gli eccessi di ottimismo, quali hanno potuto valutare e rappresentare, anche in sede di audizione, sia Bankitalia che l'Ufficio parlamentare di bilancio. In particolare, proprio Bankitalia - e spiace dover ricordare anche in questa occasione il grande convitato di pietra di questo aggiustamento di conti di ottobre, cioè il grande tema delle sofferenze bancarie e delle pesanti ripercussioni sul nostro sistema economico e quindi anche sui conti pubblici ha sottolineato come sia ormai indispensabile ridurre la spesa e concentrare le misure a sostegno della crescita; mentre l'Ufficio parlamentare di bilancio, per la prima volta dalla sua costituzione, non ha validato il quadro programmatico presentato dall'Esecutivo. Non era mai accaduto e c'è da domandarsi se siano impazziti tutti coloro che stanno valutando i numeri del Governo o se sia invece impazzito solo questo Governo. Ma per restare al tema della riduzione della spesa, tanto discussa, evocata e mai realizzata, se mai esiste, vice ministro Morando, questa è avvenuta sul previsto e non sullo *stock* accumulato. Si rende perciò evidente l'immobilità del Governo rispetto al tema della riduzione della spesa e l'assenza di tagli di carattere strutturale. Una considerazione che è avvalorata ancora una volta dai numeri, un fenomeno rilevantissimo: i circa 1,7 miliardi di tagli non più lineari, ma selettivi, previsti dalla legge di stabilità per il 2015, non sono mai stati realizzati.

una conclusione deludente dovuta alla sostanziale reintegrazione di diversi capitoli di spesa interessati avvenuta nel corso dell'esercizio. Altro che la *spending review* con cui abbiamo riempito

non è un atto altro soggetto impazzito come l'Ufficio parlamentare di bilancio o la Banca d'Italia), «una revisione attenta di quanto può o non può più essere a carico del bilancio dello Stato, in un processo di selezione della spesa non incidere negativamente sul potenziale di crescita del Paese». Sì, perché a caratterizzare la spesa corrente statale non c'è solo il dato sul personale - che, come tutti sappiamo, è incomprimibile - o quello sui consumi intermedi. peraltro è andato ben oltre le aspettative, per restare al tema che anche il vice ministro Morando prima segnalava: era prevista la riduzione del 3 per cento negli stanziamenti, mentre si è registrato l'incremento più significativo degli ultimi anni. Sulla spesa corrente dello Stato grava non poco quella per i trasferimenti alle amministrazioni territoriali, anche se, poi, ai territori viene scaricato il fardello di molti servizi e, a quei servizi, non corrispondono gli adeguati trasferimenti da parte dello Stato. un dato incombente, che dimostra come rimanga ancora irrisolta l'attuazione del federalismo fiscale; un impianto da tutti invocato, la cui completa realizzazione è continuamente rinviata ostacolata da una sovrabbondanza normativa che, però, non riesce ad affrontare adeguatamente i nodi ancora irrisolti del difficile finanziamento degli enti territoriali, della sempre sfuggente, leale collaborazione tra livelli di Governo e della responsabilizzazione fiscale degli enti territoriali. Basti pensare al marginale contributo dei Comuni all'attività di accertamento del 2015. Da ultimo vorrei ricordare un paio di questioni che considero emblematiche; anzitutto i famosi pagamenti della pubblica amministrazione. È stato provvedimento *ad hoc* per garantire alle nostre imprese di non dover più fare da banca e da finanziatori dello Stato italiano, ma poter vedere realizzato il loro onesto e giusto guadagno dopo aver fornito servizi alla pubblica amministrazione. Nonostante lo sforzo normativo e finanziario, i debiti commerciali sono diminuiti solo dello 0,3 per cento del PIL, restando a quota 65 miliardi. Chi ricorda Matteo Renzi quando, in una famosa trasmissione televisiva, dichiarava che nel giorno di San Matteo di quell'anno - correva l'anno 2014 - tutti i debiti debiti della pubblica amministrazione sarebbero stati onorati e pagati alle imprese italiane? Ecco, siamo ancora qua a fare i conti con 65 miliardi - ripeto 65 miliardi - che le imprese italiane hanno prestato allo Stato senatore Candiani)* per ciò che hanno svolto a proposito di quei consumi intermedi, cioè degli acquisti dei beni e servizi della pubblica amministrazione che lo Stato ordina, fa eseguire alle imprese, per poi non pagarle; le quali, a loro volta, non pagano i loro fornitori; i quali, a loro volta, non possono onorare i loro debiti con le banche. genera una catena, un circuito vizioso che ha portato il nostro Paese vicino al tracollo. Potrei continuare per molto ancora, signora Presidente, ma concludo, perché credo che quanto abbiamo detto sin qui da più parti sia sufficiente a dimostrare l'inadeguatezza del Governo rispetto alle sfide poste dall'ormai inderogabile necessità di risanamento della finanza pubblica; risanamento più volte declinato dallo stesso Governo nel senso del contenimento della spesa e della riduzione del debito.

ha distribuito risorse a pioggia, peraltro con risultati, dal punto di vista del riscontro dei numeri, talmente modesti da far pensare che quello spreco di denaro pubblico, raccolto dalle tasse degli italiani, sia stato distribuito

Questo è un Governo irresponsabile e sono certa che gli italiani, nel loro giudizio, ne terranno conto e, alla prima occasione che avranno, bocceranno la sua azione per aver impoverito ulteriormente il Paese, sprecato anni di congiunture internazionali che

che questo Governo nasconde ma che, evidentemente, altri si sono presi l'incarico di dimostrare: dalla Corte dei conti alla Banca d'Italia, all'Ufficio parlamentare di bilancio. Senza parlare poi degli osservatori internazionali, che ormai cominciano a non credere più alla capacità di questo Governo di portare il nostro Paese fuori da un percorso

di non verità sui numeri che il Ministro dell'economia è costretto a correggere rispetto a previsioni che definire solo ottimistiche è ancora poco. Noi voteremo contro, ricordando il nostro impegno, come quello di tutti, per migliorare i conti e la situazione economica dello Stato, sempre pronti e disponibili a trovare soluzioni, ma quelle che servono agli italiani, non quelle che servono solo a qualcuno di voi. *(Applausi noi oggi stiamo esaminando e andremo a votare il Rendiconto 2015 e l'Assestamento 2016: due anni

Se è una politica di spesa corrente - e il Governo può avere la sua valutazione - sappiamo tutti che la spesa corrente è effimera;

conti dice che per attivare la clausola di flessibilità sugli investimenti concessa per il 2016 - quindi è già stata concessa le spese di cofinanziamento non devono essere sostituite dagli investimenti finanziati interamente da risorse nazionali, così che gli investimenti pubblici totali nazionali non devono diminuire. La spesa per investimenti finali effettiva dello Stato sarebbe poi in realtà ancora più contenuta, sottraendo i pagamenti agli enti locali per specifici interventi contabilizzati anche nella spesa finale di tali soggetti.

sentito del fatto che lo Stato non ha fondi per pagare le imprese.

il Governo ci fornisca quei dati che, a suo dire, produrranno quella stima, perché altrimenti noi non potremo valutare.

Concludendo, signora Presidente, il nostro voto sarà contrario sul Rendiconto, perché ovviamente è il risultato della politica di questo Governo, e

MPL))*. Signora Presidente, colleghe, colleghi, anche quest'anno ci vengono presentati contestualmente i due disegni di legge anche se lo sforzo dei colleghi della maggioranza e del rappresentante del Governo è quello di farli passare come interventi meramente di tipo tecnico, è chiaro che hanno una portata di carattere politico.

ora siamo oltre il secondo anno di mandato e gli effetti delle politiche sbandierate dovrebbero cominciare a vedersi.

tanta stampa amica. Bene, anche questo 25 per cento di realizzazione rispetto a un montante complessivo oggi si appalesa come assolutamente insufficiente; oggi si appalesa come una ricetta che non solo non fa ripartire il Paese, non lo rilancia,

Quando si manca il centro della previsione, quando in maniera così clamorosa si manca il punto di equilibrio su cui si imposta tutta la manovra finanziaria - sapete che le previsioni per l'anno successivo si fanno sempre sulla base delle previsioni di crescita - è chiaro ed evidente - non c'è da arrampicarsi sugli specchi, cari colleghi di maggioranza - che ne discende a catena tutta

la collega del Gruppo PD ha voluto portare avanti o le argomentazioni addotte dal vice ministro Morando, perché è nella logica stessa. Non avete da giustificarvi: una volta che non avete

esaminati in Commissione. Non c'è alcun effetto positivo: non sono aumentati i prezzi, non è aumentato il consumo e non è aumentata la circolazione di denari, che consentirebbe anche

della nostra società e della nostra economia, che è rappresentato, ancora una volta, dalla stagnazione. Ad esempio, a proposito del capitolo dei pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione per le prestazioni contrattuali, quante anomalie ci sono sul versante non solo dei pagamenti, ma anche dell'azione della pubblica amministrazione. Ma quando mai fatto? Ancora una volta dobbiamo affermare che la crescita economica può essere favorita solo da scelte che diano maggiore slancio e da un programma intelligente che guardi ad una rivoluzione culturale all'interno della pubblica amministrazione, improntata a scelte giudiziose di individuazione e lotta agli sprechi, che guardi agli investimenti a medio termine e alle specificità territoriali del nostro Paese, che è così variegato, variegato, alla coesione sociale ed economica delle popolazioni dislocate nei territori e che realizzi quella necessaria parità di opportunità nell'accesso alle infrastrutture e alla mobilità dei servizi. Alla luce di queste ed altre criticità persistenti e considerato il fatto che questo è il primo dei documenti di carattere finanziario che saremo chiamati ad esaminare - si apre, infatti, la stagione della legge di stabilità

programmazione e ai numeri. Avremo modo di parlare dei fallimenti del Governo dal punto di vista della capacità di dare risposte concrete per il rilancio del nostro Paese.

un alibi per quello che ormai riteniamo un vero e proprio fallimento di tutte le previsioni economiche e finanziarie, che infatti, puntualmente, vengono smentite al ribasso. ribasso. Vogliamo stigmatizzare, inoltre, un'ulteriore attitudine del Governo che mai come in questo periodo si sta esternando, e cioè l'intento propagandistico che fa da cornice ormai alle manovre di

Anche la previsione di una crescita per il 2017 dell'1 per cento, presentata con la Nota di aggiornamento al DEF, è stata definita dal vice direttore generale di Banca d'Italia Signorini, in audizione davanti alle Commissioni bilancio di Camera e Senato, a dir poco ottimistica. Ancora più sconcertante è il fatto che il Governo leghi inesorabilmente - già dalle prime pagine - le stime di crescita e di ripresa economica del Paese nel 2017 alla vittoria del sì al *referendum* costituzionale. Nella premessa introduttiva della Nota di aggiornamento al DEF è scritto a chiare lettere, e non sto qui a ripeterlo perché il Vice Ministro lo conosce perfettamente; anzi, per la verità, mi meraviglio molto di lui. Vorremmo innanzi tutto dire non tanto sommessamente, perché confortati nel giudizio anche da moltissimi economisti, che la riforma costituzionale sottoposta a *referendum* non snellirà certamente, ma appesantirà il processo legislativo, così come farraginosamente e improvvidamente viene modificato dal testo sottoposto al giudizio dei cittadini. Per non parlare, poi, di quello che è accaduto. So quanto il Vice Ministro ha lavorato per la costituzione dell'Ufficio parlamentare di bilancio

Governo. Venendo al merito dei disegni di legge, il conto del bilancio che emerge dal Rendiconto 2015 certifica la politica fallimentare del Governo. Dal lato della spesa si evidenzia, infatti, un incremento degli impegni finali con un aumento della spesa corrente di 43 miliardi, cui ha fatto riscontro una riduzione della spesa in conto capitale, ovvero della spesa per investimenti, di ben 35 miliardi, con una flessione del 46,23 *Ad adiuvandum*, rispetto a questa tendenza distorsiva e a dispetto di tutti i proclami di Renzi sulla presunta riduzione delle tasse, si assiste nel 2015 a un aumento sia delle imposte sul patrimonio e sul reddito di 14,6 miliardi sia delle tasse e imposte sugli affari di 3,8 miliardi. Questi dati, commentati autorevolmente dal Presidente della Corte dei conti, dimostrano che abbiamo avuto ragione, noi di Sinistra italiana, quando sostenevamo che la politica di austerità a lungo andare avrebbe portato un inevitabile aumento della spesa corrente, nonostante il continuo utilizzo della *spending rewiev*; la conseguente forte riduzione della spesa per investimenti per infrastrutture e opere realmente necessarie al nostro Paese (e non ci riferiamo al resuscitato Ponte sullo Stretto di Messina); l'aumento della tassazione e la riduzione dei servizi ai cittadini, che porta con sé lo scadimento della qualità della vita, e in realtà, in generale, la depressione dal punto di vista economico del Paese. La selezione operata dal Governo nella riduzione della spesa pubblica - come sostiene il Presidente della Corte dei conti - il più delle volte è improntata a generiche e spesso contraddittorie attività di sfoltimento che non hanno interessato le cosiddette "strutture doppione" o quelle che mostrano una sostanziale mancanza di interesse pubblico, andando invece ad incidere negativamente sul personale, attraverso il blocco della contrattazione e del *turnover* che ha permesso allo Stato di risparmiare ben dieci miliardi. Senza contare, poi, molti degli interventi innescati dalla riforma Madia che devono essere portati a compimento, la cui quantificazione precisa sugli effetti finanziari è al momento impossibile. Ma per la verità abbiamo un vago sentore che anche quella, più che una riduzione, sarà un incremento delle spese stesse.

varie interrogazioni al riguardo. Istituito dalla legge n. 190 del 2014, per fare fronte a esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di un anno finanziario e che non sono prevedibili quando si approva la legge di stabilità,

sul terremoto, un forte no da parte del Governo. Riteniamo sia una domanda più che legittima e lecita, dopo il recente terremoto e la constatazione - noi più volte l'abbiamo posta all'ordine del giorno della politica - della fragilità complessiva del nostro Paese, che ci obbliga non solo a fronteggiare immediate necessità presenti nel nostro territorio, ma anche a fornire risposte di lungo respiro sul piano della messa in sicurezza delle innumerevoli fragilità territoriali ed edilizie che affliggono il nostro Paese. Ritornando al Ponte sullo Stretto, il Presidente del Consiglio, con riferimento alla sua realizzazione, ha sempre tenuto a precisare che, in ogni caso, si sarebbe dovuta dare priorità alla realizzazione delle opere veramente cruciali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese che, purtroppo, conta una altissima percentuale di opere incompiute, arrivate nel 2014 a quota 868, da 692 nel 2013, con il *record* negativo proprio della Regione Siciliana, che vede sul territorio ben 215 opere rimaste al palo. opere rimaste al palo. Al netto di ciò che noi abbiamo sempre sostenuto, riteniamo comunque inammissibile che il Presidente del Consiglio, dopo il disastro di Genova, il disastro ferroviario in Puglia e il drammatico sisma dello scorso 24 agosto, rilanci la realizzazione, per meri scopi pre-elettorali, di un'opera assurda, inutile e dannosa come il ponte, tra l'altro in una delle aree territoriali più sismiche del Paese.

un maggior sostegno per le non autosufficienze; un impegno aggiuntivo sul rimborso dei medicinali innovativi; un intervento finalmente decisivo contro il rischio sismico e idrogeologico; un intervento forte sul sistema territoriale dei servizi socio-educativi,

la questione riguardante il trasporto pubblico, il trasporto su ferro. Non ci sono mai state date risposte significative. Ma quello che si evince, proprio nel momento in cui abbiamo

del Governo. Quindi, voteremo molto convintamente contro il Rendiconto e contro l'Assestamento, perché abbiamo una visione concreta

ed assolutamente irresponsabile continuare a giocare con i numeri e fare previsioni che già si sa in partenza che saranno puntualmente smentite dai fatti, mentre non si fa invece invece assolutamente nulla per mettere in atto politiche diverse, che possano dare davvero un futuro al nostro Paese. Non sarà la riforma costituzionale a dare un futuro all'Italia; un futuro all'Italia potranno darlo soltanto politiche serie di investimenti per un vero *green new deal*, che può portare il Paese fuori dallo stallo e dalla grave crisi economica. Signora Presidente, onorevoli colleghi, all'ordine del giorno sono posti passaggi di grande rilevanza nel ciclo di bilancio, passaggi attraverso i quali vengono presentati alle Camere i risultati definitivi

Dall'analisi, per quanto sommaria, dei saldi di bilancio dello Stato per il 2015 si evince in prima battuta un complessivo miglioramento rispetto alle previsioni definitive per la maggior parte dei parametri, anche rispetto ai risultati consuntivi del 2014.

dopo tre anni di decrescita (meno 2,8 nel 2012, meno 1,7 nel 2013, meno 0,3 nel 2014) ritorniamo finalmente in territorio positivo. Certamente non è molto, specie se si considerano le attese di gran parte dei nostri cittadini; ma è un inizio da cui partire per rafforzare l'azione di Governo. Nel Rendiconto 2015 ci sono due indicatori significativi: il saldo netto da finanziare è pari a 41,5 miliardi e il ricorso al mercato è pari è pari a 257 miliardi. Sono valori nettamente migliorativi rispetto alle previsioni iniziali e a quelle assestate, oltre ad essere più favorevoli rispetto ai risultati del 2014, risultando, oltre al resto, nettamente al di sotto dei tetti massimi stabiliti dalla legge di stabilità per il 2015. risultati positivi, che ci hanno permesso di chiudere il 2015 con un rapporto *deficit*-PIL pari al 2,6 per cento, un risultato decisamente migliore rispetto al triennio precedente, che pure aveva visto l'indebitamento posizionarsi costantemente intorno al limite del 3 La politica economica messa in campo dal Governo dimostra quindi di funzionare e di dare risultati positivi, per quanto ancora quantitativamente modesti, anche se certamente i problemi da risolvere restano ancora molti, ad iniziare da un debito pubblico importante che, nonostante i tanti sforzi compiuti, si continua a far fatica a ridurre. La legge di stabilità per il 2015, i cui effetti sono ricompresi nel Rendiconto dello Stato che oggi analizziamo, così come anche quella relativa al 2016, hanno costituito dei tasselli di fondamentale importanza nell'ambito dell'azione organica complessiva che il Governo deve attuare per sostenere la ripresa economica. La strategia è favorire la crescita e l'occupazione, realizzando riforme strutturali ormai non più posticipabili. Ricordo solo la riduzione dell'IRAP a carico dell'impresa con l'esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro per i dipendenti a tempo indeterminato, che ha segnato un passo importante nel processo di alleggerimento del cuneo fiscale; gli sgravi contributivi relativi alle nuove assunzioni riconfermati nell'anno successivo, seppure per importi più limitati, hanno costituito, insieme con le novità introdotte dal *jobs act*, una spinta per la nuova occupazione. È proprio di ieri la rilevazione dell'ISTAT che certifica 439.000 occupati in più nel periodo luglio 2015-luglio 2016. Le molte misure finalizzate a stimolare gli investimenti e le innovazioni aziendali, il rifinanziamento della legge Sabatini, il credito di imposta per spese di ricerca e sviluppo, il nuovo regime di *patent box* hanno promosso e sostenuto la crescita delle nostre aziende, perché il reddito prima di essere redistribuito deve A quanto già detto si deve poi aggiungere la legge delega per la riforma della pubblica amministrazione e la riforma della scuola. Certo, tutto questo non basta, come dimostra la discussione già avviata sulla Nota di aggiornamento del DEF; documento, quest'ultimo, che mostra chiaro scuri su cui dovremmo riflettere attentamente. Non si può sfuggire all'impressione che troppo spesso il Governo sia frenato da una discussione non sempre serena all'interno del partito di maggioranza, le cui fratture finiscono per ritardare l'azione amministrativa e quindi l'efficacia delle misure prese sull'andamento effettivo dell'economia nazionale. Ci rincresce il fatto di dover rilevare come gli investimenti, sia pubblici che privati, stentino a svilupparsi, mentre cresce la spesa corrente al netto degli interessi, e che alcune misure prese, come il *bonus* di 80 euro, non abbiano prodotto i risultati sperati in termini di crescita della domanda interna e quindi di sviluppo. C'è, pertanto, di che lavorare. Siamo convinti che il Paese intero si attenda da parte di tutte le forze politiche italiane una coesione maggiore, come più volte auspicato dal nostro presidente Mattarella. è, infatti, l'elemento essenziale che determina un orizzonte favorevole allo sviluppo, dando maggiore certezza agli operatori; quella serenità che spinge le famiglie italiane a consumare, gli imprenditori a investire e gli apparati amministrativi dello Stato e degli enti locali a prodigarsi per dare ai propri cittadini servizi migliori e più efficienti. Come si sa, signora Presidente, AL-A persegue da tempo quest'obiettivo, con un'ostinazione che non demorde nemmeno di fronte alle valutazioni, molto spesso ingiuste, di una stampa non proprio oggettiva e incapace di scorgere, di là delle alchimie parlamentari, il segno più profondo di una nostra presenza. Le scelte finora compiute non vanno nella direzione della lottizzazione politica, ma sono, al contrario, frutto della lucida consapevolezza delle gravi difficoltà che il Paese deve ancora affrontare e che non si risolvono né con la politica del "vaffa", né con l'opposizione pregiudiziale, ma con un confronto sereno, capace di valorizzare quel che c'è di buono nell'azione del Governo. Ma siamo anche pronti alla critica, quando riteniamo quell'azione si dimostra insufficiente. Voteremo pertanto a favore, e non perché non abbiamo osservazioni da fare, che svilupperemo coerentemente nell'imminente sessione di bilancio, ma perché le luci prevalgono sulle ombre e perché i documenti al nostro esame sono testimoni di uno sforzo autentico, seppure per il momento insufficiente.

non si è ancora pienamente divincolato dai tentacoli della crisi economica. I principali indicatori di finanza pubblica, tuttavia, mostrano segnali di ottima tenuta e danno il segno di conti pubblici in ordine e in miglioramento. Nello specifico del disegno di legge, ad esempio, il Fondo esigenze indifferibili, inizialmente dotato di 25 milioni di euro, viene incrementato sino a 955 milioni di euro: lungi dal rappresentare un assegno in bianco alla Presidenza del Consiglio, il meccanismo di funzionamento del Fondo prevede l'individuazione delle destinazioni tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che sarà ovviamente oggetto di scrutinio consultivo parlamentare, in modo da garantirne un utilizzo trasparente ed efficiente. D'altronde, proprio il vice ministro Morando ci ha fornito delucidazioni in Commissione circa le modalità di utilizzo di tali risorse, che non possono essere impiegate per fini prestabiliti dal Governo e non resi noti al Parlamento. Vorrei brevemente parlare della revisione della spesa. Ritengo che uno dei capitoli principali che assicura la tenuta dei conti pubblici sia stato negli ultimi anni la riforma pensionistica: l'onere pensionistico è stato reso completamente sostenibile anche nel lungo periodo, intervenendo nel contempo a tutela delle persone ingiustamente penalizzate nel proprio assegno mensile. In questo specifico settore, si deve mantenere tale approccio, relativo alla razionalizzazione della spesa pensionistica, garantendo forme di maggiore equità sociale e l'astensione da interventi che possano intaccare la pensione dei cittadini. Altro tema, che rientra a pieno titolo nella *spending review*, è quello legato agli acquisti di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione, su cui pure si sono registrati miglioramenti degni di nota. Anche le risorse destinate al pubblico impiego hanno rappresentato una voce di bilancio virtuosa grazie agli sforzi fatti da questo Governo e dai precedenti. Le testimonianze di un effettivo processo di riordino della spesa sono rintracciabili anche nei numeri di un significativo avanzo primario. Relativamente alla prossima manovra di bilancio, ormai vicina, auspico un confronto serio e sereno che, nell'ambito di un rigoroso rispetto dei regolamenti europei, garantisca una manovra il più espansiva possibile, al fine di garantire spazio alla ripresa del sistema economico. Presidente, concludo augurandomi che si possano introdurre politiche per la crescita più strutturali e meno episodiche rispetto al passato, citando l'esempio dell'eventuale fiscalizzazione degli oneri contributivi su scala triennale, con evidente beneficio per la programmazione degli investimenti privati.

- 9 miliardi di risparmio pubblico. Questi soldi servirebbero a fare quegli investimenti di cui il nostro Paese ha veramente bisogno. Questi soldi servirebbero finalmente ad alimentare quell'indice, che è il PIL,

Cos'è cambiato rispetto ai dati mortificanti di questo Rendiconto? Perché mai dovrebbe esserci questa crescita? È dovuta forse alle riforme strutturali?

spartirsi di nuovo i rimborsi (perché niente verrà eliminato), con sì e no 50 milioni di risparmio? Questa sarebbe la grande riforma strutturale? Il punto su cui vorrei soffermarmi è soprattutto quanto ha detto il Padoan. Voi avete previsto le clausole di salvaguardia, dovute a quell'immane errore che sono stati gli 80 euro, che stiamo pagando ancora. Quelle clausole di salvaguardia le avete messe voi,

cosa avete fatto con la decontribuzione?

Avete appesantito il cuneo fiscale di un miliardo! Questa è la sacrosanta verità, perché quando non ci sarà più questa manovra *spot* il cuneo fiscale resterà più pesante per un miliardo. Questo bisogna dire alle imprese, perché è la verità. Non Non prendiamoci in giro dicendo che, in realtà, vogliamo alleggerire il cuneo fiscale, perché lo abbiamo appesantito. E non mi dite della componente lavoro dell'IRAP, perché lo sapete bene che per molte delle piccole e medie imprese, soprattutto quelle del Sud, per un serie di meccanismi fiscali, questa non era assolutamente dovuta. Voi avete fatto una *spending* *review* andando proprio sulla parte produttiva, andando proprio su quelle imprese, soprattutto le artigiane, che andavano a risolvere un problema annoso quale la disoccupazione di lunga durata. E in agosto, che è un mese in cui - come si sa - storicamente si assume di più, non siete neanche riusciti a recuperare la perdita dei 63.000 posti di lavoro di luglio. Questo bisognerebbe dire e valutare cambiando politica economica, cosa che invece non si fa assolutamente. la *spending review*, noi siamo favorevoli, ma non mi potete dire che è stata fatta veramente in maniera puntuale, né mi potete dire che verrà dalla pubblica amministrazione o addirittura dalla legge di contabilità. Quando non è riuscito a fermarvi neanche l'articolo 81 della Costituzione a fare nuovo debito pubblico, voi mi dite che la legge di contabilità vi fermerà? Chiedete sforamenti su sforamenti e lo faremo anche nel prossimo aggiornamento del DEF. Che cosa dovrebbe mai bloccare la legge di contabilità,

previsto un taglio di 4 miliardi di euro a carico delle Regioni, di cui 3,5 a carico della sanità. Lo avete messo voi nero su bianco. Nel 2018 ce ne saranno altri 5, di cui 4,5 miliardi a carico della sanità. Dite che nei vostri documenti di programmazione prevedete che la spesa pubblica deve diminuire a carico delle amministrazioni locali ma non del Governo centrale, che si mantiene le mani libere per dare i *bonus*,

quindi uno scarto dello 0,4 per cento; ora quello scarto tra la nostra disoccupazione e la media europea è arrivato all'1,5 per cento. Stiamo diventando altro che la locomotiva d'Europa: il carro, la ruota di scorta dell'Europa. Noi questo

perché tutto quello che avete fatto, lo avete certificato voi in questo documento; è stato assolutamente sbagliato e oltremodo dannoso. Quindi gloria, evviva i nostri no! Peccato che non li abbiate colti e peccato che continuiate a non voler cogliere la nostra programmazione per questo Paese. il vantaggio della discussione sul bilancio di Assestamento e sul Rendiconto è duplice quest'anno. Il primo è quello di sempre: preferisco misurarmi sempre non su scenari, ma su previsioni a date così brevi, come l'Assestamento, che hanno un grado di attendibilità quasi vicino alla certezza, giusto per il brevissimo periodo che separa la previsione in assestamento dalla conclusione dell'anno e, quindi, dal bilancio definitivo. Si ha dunque una rappresentazione dello Stato e della finanza pubblica, ravvicinata, attendibile e molto molto vicina alla certezza. Il secondo vantaggio quest'anno è che, siccome quest'oggi si inizia in Commissione bilancio la discussione sulla Nota di aggiornamento del DEF, sarà quella la sede in cui si discuterà sugli scenari e quindi oggi ci possiamo concentrare invece, non su questo tipo di orizzonte, ma sull'orizzonte previsivo a breve termine del bilancio di assestamento. Pertanto sono esentato oggi dal fare i ragionamenti sugli scenari. Se guardiamo allora il bilancio di Assestamento, direi che l'unica cosa cui può essere avvicinato è una sorta di bollettino delle perdite. Se lo guardiamo in termini di competenza, il disegno di legge di assestamento evidenzia un peggioramento del saldo netto da finanziare, del risparmio pubblico e dell'avanzo primario. Ma siccome io sono più legato alle previsioni di cassa, perché il nostro grande problema è il debito e alla fine il debito è molto più comparabile in termini di cassa, cerco di vedere previsioni assestate per la cassa. Peggio: tutti saldi peggiorano con entità significative. Pensate che il saldo netto da finanziare passa da 98,1 miliardi a 107 miliardi il risparmio pubblico passa da -59,3 a -61 miliardi di euro (il risparmio in cifre negative è ovviamente un peggioramento); la necessità di ricorrere al mercato - dato importante - registra un incremento di 9,3 miliardi, raggiungendo l'importo di 330 miliardi l'avanzo primario, partendo da un valore di -14 miliardi giunge ad un importo di -27 miliardi di euro. Questo è lo stato delle finanze pubbliche italiane. Non c'è un solo parametro in questo momento che ci conforti. Lasciamo perdere le cose complesse (ce ne occuperemo in altra sede): queste sono cose piuttosto semplici e indicano un peggioramento di tutti i parametri vitali della finanza pubblica.

disponendo che la quantificazione dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici sia portato a 64 miliardi rispetto a 53,4 miliardi euro. Non mi nascondo che ci sono anche questioni tecniche quando si tratta di simili grandezze, ma in un contesto come quello in cui stiamo vivendo questi giorni, dire che comunque è possibile che lo Stato ricorra di più all'emissione di titoli e quindi all'indebitamento non è un segnale positivo, e questo ovviamente ha un grande rilievo nella nostra decisione parlamentare.

uno dei parametri che va bene. Pensate alla questione del debito. Da sempre abbiamo detto: quest'anno va un po' meglio. No, il debito

È possibile derogare a vincoli pattizi se si fa un investimento sul futuro e si spende per investimenti. Invece no:

la convinzione che l'operato di questo Governo, non solo non sta risolvendo i problemi della finanza pubblica italiani, ma - anzi

consentire un miglioramento della spesa in conto capitale e, per questa via, si possono chiedere deroghe ai vincoli pattizi per l'investimento sul futuro.

poi anche quelle istituzionali. Certo, una qualche relazione tra le due riforme c'è, ma non è detto - e a questo punto, non è vero - che alcune riforme

perché riteniamo che i dati confermino la correttezza di una linea di politica economica e sociale perseguita in questi anni.

anche l'occupazione è tornata a vedere il segno positivo; nello stesso tempo, siamo riusciti a tenere sotto controllo la spesa e a invertire la tendenza anche sulla pressione fiscale. Questi sono i dati sintetici. Abbiamo fatto tutto ciò in una condizione molto difficile, che a me piace paragonare

il precipizio della recessione e a sinistra quello del *default*, della crisi del debito, dell'insolvenza dello Stato. Noi dobbiamo camminare su questo crinale molto stretto e molto difficile. Onestamente in quest'Aula, al di là di tante piccole critiche di merito, sulle quali tornerò e che hanno tutto il diritto di essere prese in seria considerazione, dal punto di vista della strategia generale ho sentito solo qualche invito a buttarsi in un precipizio oppure nell'altro. C'è una parte che dice che dobbiamo

il pareggio di bilancio strutturale è un feticcio, sfondiamo il 3 per cento come fanno altri Paesi e vedremo che la crescita riprende. Questo è l'invito a buttarsi nel precipizio opposto, cioè a tornare a rendere inaffidabile il nostro Paese sui mercati (e sappiamo che ogni anno dobbiamo vendere centinaia di miliardi di debito), tornare con lo *spread* al 5 per cento, dove ci siamo trovati all'inizio di questa vicenda, in una situazione finanziaria drammatica che poi metterebbe rapidamente in discussione qualunque obiettivo di crescita.

è un percorso sul quale il Governo italiano è fortemente impegnato: abbiamo infatti bisogno che, accanto al lavoro di risanamento, che è necessario venga fatto dagli Stati nazionali,

federazione di Stati, che mantengono ancora una forte sovranità sulle politiche economiche e nello stesso tempo vogliono avere in tasca la stessa moneta), accanto a questo elemento di disciplina ci sia un motore espansivo che si accenda a livello federale. Quando il nostro Presidente del Consiglio invita a fare come in America, intende esattamente questo. Negli Stati Uniti d'America gli Stati che compongono

c'è il motore federale che si accende e c'è un'enorme spinta alla crescita, dovuta al fatto che l'azione del Governo federale e il Tesoro americano favoriscono

che è quella che ci tiene in vita in questo momento. Ho ascoltato, come sempre con attenzione, le parole del senatore Azzollini: se ci togliamo questo ossigeno, soffochiamo. Altro è dire che questo ossigeno, quel poco che c'è, va usato in maniera intelligente. Qui le parole chiave sono due: una è la parola «riforme», l'altra è la parola «investimenti».

Fuor di metafora vuol dire che gli 800 miliardi di euro di spesa pubblica devono essere riqualificati, posto che non possono crescere, ma semmai devono diminuire un po'. Per farli diminuire un po' e produrre crescita e uguaglianza sociale, li dobbiamo riqualificare, ristrutturando la spesa pubblica, attraverso le riforme, cominciando dall'alto, ovvero dal Parlamento. Se infatti il Parlamento non funziona, non funziona lo Stato e, se non funziona lo Stato, l'economia va a farsi benedire.

volta ha detto che, senza conoscere il contenuto della manovra, non può validare l'obiettivo di crescita dell'1 per cento. Questo è quanto ha detto l'UPB.

penso che intanto noi tutti dobbiamo essere contenti del fatto che si è aperta una discussione di merito a partire da dati certi. Questo è il merito principale di aver costituito l'Ufficio parlamentare di bilancio. Mi fa piacere che oggi l'Assemblea, e in particolare le opposizioni, plaudano a scena aperta al fatto che abbiamo finalmente un'autorità indipendente che certifica il bilancio. Ebbene, questo è quello che abbiamo voluto quando abbiamo varato il nuovo articolo 81 della Costituzione: avere un'autorità indipendente che certifichi il bilancio e che introduca un elemento di dialettica concreta, concreta, realistica e non ideologica nel nostro confronto. Il problema, adesso, è che possiamo chiudere la contraddizione in due modi, e concludo, signora Presidente. Il primo è quello che ci ha chiesto ieri

L'altra strada per chiudere la contraddizione è dire che dobbiamo fare una manovra che renda realistico l'obiettivo dell'1 e la maggioranza con lui - è che noi renderemo realistico questo obiettivo. Faremo crescita e faremo occupazione dentro il quadro di competitività europeo.

che questo passaggio sorprendente della settimana scorsa era stato determinato da una inversione dell'ordine del giorno richiesta il giorno dopo che il Governo autorizzò l'apposizione della fiducia sul testo uscito dalla Commissione; fiducia che poi non è mai stata posta e che, comunque, determinò l'inversione dell'ordine del giorno e l'esame del Ora, mi chiedo, a distanza di una settimana, se le diatribe e le contese che si erano aperte all'interno della maggioranza non si siano concluse perché, a questo punto, credo che ci troviamo di fronte a una grande difficoltà:

se non sia più serio affrontare il provvedimento; nel caso, richiedere un ritorno in Commissione dove finalmente il ministro Orlando chiarirà se la questione debba andare in un senso piuttosto che in un altro. È però ora di finirla con questo modo di lavorare in Senato o, meglio, di non lavorare. È evidente che in questo momento, alla luce del voto del 4 dicembre, nessuno vuole affrontare qualunque tipo di argomento comporti un coinvolgimento. Si parla del processo? No, è troppo divisivo e non lo si vuole affrontare. C'è il disegno di legge sulla concorrenza? No, anche quello è divisivo e, quindi, non possiamo toccare neanche quello.

dobbiamo, proprio per assecondare la volontà del Governo, non fare più niente, per dare l'idea che il Senato sia un ente inutile e quindi debba essere abolito votando sì al *referendum*. Perché questa è la volontà. *(Applausi dai

Presidente della Repubblica, che ha definito indegno il Parlamento e, quindi, anche questo Senato: indegni saranno sua sorella e suo fratello, non certo il Senato! Signora Presidente, invito il collega Calderoli, del quale conosciamo l'attenzione istituzionale, a rivolgersi

che io credo siamo in condizioni di concludere a brevissimo. Quindi il mio intervento è semplicemente per ribadire la mia speranza che l'intenzione della maggioranza

La mia è una proposta molto semplice. Sappiamo benissimo che anche i *set* cinematografici e le produzioni costituiscono un importante volano di promozione dei territori.

propongo che ci sia una quota di riserva per le produzioni nel Mezzogiorno, in maniera tale da incentivare i produttori a recarsi in quei territori, come già peraltro in parte accade. È necessario tuttavia aumentare sempre più la loro presenza in quei territori, anche e soprattutto al fine di agevolarne uno sviluppo economico assolutamente coerente con i tempi e con le potenzialità dei

che tocca un argomento sul quale a lungo si è dibattuto in Commissione, ovvero i criteri di erogazione dei fondi e dei finanziamenti al comparto cinematografico. Sappiamo che uno degli aspetti innovativi di questo disegno di legge è il passaggio da un sistema di erogazione dei contributi di tipo selettivo a un sistema di tipo misto, selettivo e automatico. In questo passaggio, però - a nostro avviso nel disegno di legge presentato dal ministro Franceschini, quello oggi in esame nel testo uscito dalla Commissione, la proporzione tra contributi selettivi (dati in base alla qualità culturale dell'opera

intervenuta una qualche realtà cinematografica potente, che probabilmente ha come Presidente qualcuno che ha dei legami familiari anche con qualche Ministro di questo Governo: tutte ipotesi, non si sa, ma è possibile che vi sia stato un intervento) la volontà emendativa di portare i contributi selettivi al 25

affinché riprendano in considerazione la proposta emendativa della relatrice Di Giorgi che bene aveva compreso che la percentuale dei contributi selettivi dovesse essere aumentata al 25

per fare un favore al Movimento 5 Stelle, ma per ascoltare i tanti operatori del mondo del cinema che, a gran voce e in ripetute occasioni, hanno chiesto alla relatrice e al Governo di riflettere su questo punto e di concedere questa percentuale.

sprovviste di sistema di controllo marcia treno (SCMT) e gestite dalle Ferrovie del Sud Est, a seguito del disastro ferroviario del luglio scorso, vige il limite di velocità di 50 chilometri così come imposto e previsto dall'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria. Signora Presidente, sappiamo come il diritto alla sicurezza debba andare di pari passo con il diritto alla mobilità. alla mobilità. Ferrovie del Sud Est, di cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è socio unico, non è in grado di garantire la mobilità in modo autentico e, soprattutto, decente. La riprogrammazione degli orari dei treni, in ragione del nuovo limite di velocità, vede un prolungamento della durata dei transiti da un minimo

del Sud Est è imputata la gestione delle tratte operate con i pullman. Sono settimane ormai che studenti, soprattutto di Campi Salentina e del Nord Salento, non riescono ad arrivare a scuola in orario. Più volte gli utenti non solo non vengono fatti salire, ma addirittura vengono fatti scendere dalle vetture per questioni di sicurezza. ha fatto il giro dei *social* la foto, pubblicata successivamente anche da quotidiani locali, di diversi ragazzi seduti negli alloggi dei bagagli, perché lo spazio era saturo di passeggeri. Chiedo quindi, attraverso questo mio intervento, al ministro Delrio e a lei, Presidente, perché si faccia latore di questa mia richiesta, di venire a riferire in quest'Assemblea se esiste un piano di sviluppo e di ammodernamento delle linee gestite da Ferrovie del Sud Est e se, quindi, il Ministero si sta adoperando per allineare gli *standard* della mobilità della Regione pugliese, sia su binario che su gomma, a quelli delle altre Regioni del nostro Paese.

e la più grande realizzazione era dar loro sicurezza e un tetto dove poter vivere serenamente. Poi i problemi che ormai conosciamo bene: la crisi finanziaria, i clienti che non pagano. Le difficoltà aumentano e si entra dentro a un vortice di angoscia e disperazione. Fino a quando arriva il fisco, percepito come un mostro, a portarti il conto, non riconoscendoti l'onorabilità nei pagamenti avuta fino a poco prima, non valutando la tua condizione di sopravvivenza e dignità. Il fisco vuole tutto e velocemente. Giuseppe, ma potrebbe chiamarsi con altri mille nomi, si è consumato negli anni; le cartelle di Equitalia aumentavano in modo esponenziale, era impossibile poter restituire solamente attraverso il sudore della propria fronte. Da lì l'odissea del pignoramento della sua unica casa, costruita mattone su mattone. Aveva bussato alle banche per essere aiutato: niente da fare. Le banche continuano a tener chiusi i rubinetti per i cittadini comuni, nonostante il Governo abbia varato provvedimenti in favore delle banche per rimettere in moto l'economia italiana. Non è servito a nulla. Le piccole medie imprese non le aiuta nessuno, gli istituti di credito danno i soldi alle grandi imprese Come parlamentari abbiamo il dovere di cambiare le leggi che strozzano il cittadino comune. Bisogna varare una riforma vera del fisco e della riscossione, che renda sopportabili gli alti livelli di tassazione e che metta tutti in condizioni di poter eventualmente ripagare i propri debiti, senza portare le persone in mezzo a una strada, alla disperazione o al suicidio. Venerdì il piccolo imprenditore non ce l'ha fatta; dopo che la casa è stata venduta all'asta ha fatto il gesto estremo: si è tolto la vita. Giuseppe era un concittadino della senatrice Laura Bottici e mio, persona buona e stimata di Carrara, che giustificava chi non lo pagava, perché diceva alla moglie Antonella: «cosa vuoi, non mi paga perché anche lui non riesce a mandare avanti la famiglia». Questi sono i veri imprenditori italiani, solidali e di coscienza, e spesso ricevono trattamenti vessatori da parte di uno Stato cieco e sordo ai veri bisogni delle persone. Oggi chi si uccide per problemi economici conta il 45 per cento tra gli imprenditori e il 42 per cento tra i disoccupati. Diciamolo ad alta voce: il fisco è forte con i deboli e debole con i forti. Ma chi è il responsabile di tali scelte? Siamo noi. Noi legislatori che indirizziamo le politiche e le scelte. Non possiamo permettere allo Stato e a Equitalia di togliere la speranza ai cittadini. Il Movimento 5 Stelle si è sempre battuto e continuerà a battersi per garantire a tutti un tetto sicuro, un reddito un reddito di cittadinanza e leggi umane. Desideriamo ardentemente che lo Stato sia percepito come una grande madre, che nel bisogno c'è e protegge dignitosamente i suoi cittadini come figli, ognuno prezioso nella propria singolarità.

in collaborazione con il dipartimento di epidemiologia del Servizio sanitario del Lazio, della ASL di Taranto, di ARPA Puglia e di Ares Puglia. E se ne chiede ancora vidimazione scientifica al ministro Lorenzin. Ebbene, questo rilevante e autorevole studio mette nero su bianco una relazione di causa-effetto tra le emissioni industriali del complesso ILVA e il danno sanitario riscontrato. Sono state coinvolte in questo studio oltre 321.000 persone, in un considerevole lasso di tempo. Gli inquinanti scelti come traccianti sono il PM10 e l'SO2, ossia le polveri sottili e l'anidride solforosa. Sono risultati responsabili di nuovi casi di tumore al polmone per un più 29 per cento per le polveri e per un più 42 per cento per l'anidride solforosa. È allarme sanitario. Questo è il risultato di dieci decreti ILVA, dal 2012 ad oggi; questo è il risultato di aver voluto irresponsabilmente scavalcare il sequestro della magistratura di oltre quattro anni fa, a colpi di decreto.

Signora Presidente, voglio affrontare due terribili fatti che le cronache di Roma e di Asti, ieri e oggi ci hanno raccontato. Due terribili storie che riguardano due minori; a Roma, quella del bambino di undici anni, annegato nel canale di irrigazione a Maccarese, su cui la procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo. Un articolo del «Corriere della Sera» ci racconta infatti una storia tristissima. Risulta che agli psicologi, agli insegnanti di sostegno e agli assistenti messi a disposizione dal Comune di Fiumicino, il bambino aveva raccontato di essere stato picchiato, di vari maltrattamenti e alcuni mesi fa, davanti agli insegnanti di sostegno, era scoppiato in lacrime, in un pianto disperato dicendo: «mi sono stufato di questa vita, ora mi ammazzo. A scuola non ci voglio più andare perché qui tutti ce l'hanno con me e mi prendono in giro».

Risulta maltrattata dal padre e dalla madre, minacciata di morte, lasciata senza cibo e terrorizzata. Gli investigatori, che dopo le segnalazioni della scuola sono intervenuti con indagini ambientali, l'hanno definita una Cenerentola. Infatti alla sorellastra coetanea venivano comprati vestiti e giocattoli e veniva nutrita con il cibo migliore. A lei nulla, solo botte e frasi del tipo «ti portiamo nel bosco e ti facciamo mangiare dai lupi e dai cinghiali» oppure «ti buttiamo nell'immondizia». I genitori sono stati arrestati e le due bambine affidate ai servizi sociali. Sembrano due notizie di cronaca, due eventi isolati, ma non sono casi eccezionali e sarebbe sbagliato se pensassimo

anche importanti. Serve che l'Italia si doti, ovunque e comunque, di servizi presso i quali questi ragazzi infelici, con problemi di maltrattamento, possano trovare accoglienza.

frutto di collaborazione con esperti del settore dei maltrattamenti e degli abusi sui minori, aveva sottolineato la necessità di intervenire con immediate assicurazioni di tutela, ma anche con l'ascolto e con l'attenzione psicoterapeutica necessaria per l'elaborazione del trauma a cui questi minori sono sottratti. In Italia abbiamo leggi dure contro l'abuso e il maltrattamento, ma non abbiamo - come dicevo prima - un'adeguata rete di servizi in grado di curare e tutelare i bambini e i ragazzi abusati.

corretto il tiro e ha avviato un importante cambio di passo sui minori. Basti pensare allo specifico intervento contro la povertà educativa e materiale, con specifico finanziamento, ad altre misure importanti a sostegno della genitorialità. Occorre però proseguire su questa strada e rafforzarla, anche attraverso il potenziamento della rete dei servizi. Lo dico in modo molto chiaro: occorre scegliere e sostenere, insieme ai singoli interventi, il rafforzamento della rete di servizi per il sostegno alla genitorialità e creare servizi capaci di accogliere, curare e tutelare i minori maltrattati ed abusati; servizi e in rete dunque, e una capacità programmatoria per l'integrazione, che vada dalle scuole all'integrazione sociosanitaria, in grado di lavorare complessivamente sulla genitorialità, sul sostegno, quindi anche sulla prevenzione, e successivamente anche sulla presa in carico. Questo - come ho detto prima - riguarda in modo particolare le Regioni che hanno ancora oggi una totale autonomia e competenze sociali occorre che le Regioni stesse mettano al centro della loro attività questo tema. Alle Regioni che hanno buone prassi chiedo di avere uno scatto d'orgoglio e dare visibilità ai loro lavori, anche perché le buone prassi servono per poter

curare e tutelare i minori dai maltrattamenti e dagli abusi necessiti della continuità della presa in carico, e la continuità è data in primo luogo dalla stabilità del personale.

lillipuziano sindacato di Polizia sempre a caccia di nuovi iscritti, per voce del segretario Maccari. Sinceramente non so chi sia Maccari, lo conosco solo dalla cronaca locale veneta, dove si legge che probabilmente ha fatto fermare un treno su cui viaggiava in una stazione dove non doveva fermarsi, per poter scendere, spendendo la sua figura di incaricato sindacale, con gli agenti della Polizia ferroviaria. Detto questo, non posso che esprimere profondo stupore per la relazione dei periti nominati dal Le ecchimosi sul corpo di Cucchi da cosa derivano? Come si sono formate? Sono un chiaro segno di pestaggio, indegno per rappresentanti dello Stato. Sicuramente quelle ecchimosi non sono segno di un attacco epilettico. alle "mele marce" nelle Forze dell'ordine: lo dobbiamo a chi, con la divisa, opera per il bene del cittadino e della legalità. Si faccia pulizia tra le Forze dell'ordine, si approvi il codice identificativo delle divise e si faccia giustizia.

Porto, infine, solidarietà a Ilaria e all'intera famiglia Cucchi per l'ennesimo schiaffo al loro e al nostro dolore.

in modo che risulti sostenibile solo a patto di curare una minoranza dei malati. In questo modo si ingiunge un razionamento senza precedenti, che non solo viola l'uguaglianza davanti alla salute, ma costringe a usare i farmaci nei malati più gravi, che ne possono trarre poco beneficio, e ad aspettare che si aggravino quelli che potrebbero evitare i danni irreversibili al fegato. Non è un effetto indesiderato, ma voluto. I Governi che vorrebbero usare la flessibilità prevista dai trattati internazionali per garantire l'accesso a farmaci essenziali, ma troppo costosi, si trovano spesso minacciati da indebite pressioni di natura politica o economica da parte di altri Stati o imprese multinazionali, nel Rapporto sull'accesso ai medicinali, prodotto da un *panel* di esperti incaricati dal Segretario generale delle Nazioni Unite e pubblicato il 14 settembre scorso. La divaricazione tra il modello d'innovazione guidato dal profitto e le priorità del diritto alla salute è arrivata al limite di rottura, come riportato dalla rivista britannica «The Lancet», che a proposito titola: «Lo *status quo* non è più un'opzione». In altre parole, così non possiamo può andare avanti. Ma si potrà andare avanti con le licenze obbligatorie anche in Paesi ricchi come l'Italia? Ciò sembra difficile se non si trova il modo di modificare gli attuali rapporti di potere che consentono alle multinazionali e alle maggiori potenze (Stati Uniti in testa) di bloccare sul nascere ogni tentativo di usare i margini di flessibilità degli accordi commerciali per garantire il diritto alla salute. Tutto il nodo sta nei brevetti: nati per tutelare i diritti intellettuali dei ricercatori e incoraggiare l'innovazione, si sono ormai trasformati in una semplice leva finanziaria. Il caso del Sofosbuvir non è unico, ma esemplare anche da questo punto di vista. I brevetti sviluppati da piccole imprese sono poi ceduti a importi che non hanno alcun nesso con i costi di ricerca e sviluppo già sostenuti, ma appaiono calcolati sulla base dei profitti che si possono prevedere. Il risultato è disastroso sul piano sia dell'efficienza sia dell'equità. il prezzo dei nuovi farmaci antiepatite C è imposto, per ogni Paese, al livello più alto possibile per la ricchezza nazionale, in modo che risulti sostenibile solo a patto di curare una minoranza dei malati. In questo modo si ingiunge un razionamento senza precedenti, che non solo viola l'uguaglianza davanti alla salute, ma costringe a usare i farmaci nei malati più gravi, che ne possono trarre poco beneficio, e ad aspettare che si aggravino quelli che potrebbero evitare i danni irreversibili al fegato. Questo - secondo me - non è un effetto indesiderato, ma voluto. cosiddetti *delinked*, in realtà sono già svincolati da qualsiasi ragionevole punto di riferimento e sarà difficile fare marcia indietro senza rivedere tutta la logica del dominio del profitto nelle attività della salute. È per questo motivo che vi invito a firmare e soprattutto a portare in discussione la mia mozione. Sarà forse un meccanismo un po' complesso, forse anche un po' troppo semplice, forse anche una furbata, come qualcuno ha detto, ma è un modo per sganciarsi da questo meccanismo basato solo ed esclusivamente sul profitto e non sulla salute della popolazione.

ma ad oggi non ci sono provvedimenti relativi alla ricostruzione. Il 1° settembre il ministro Padoan ha adottato un decreto ministeriale per la sospensione dei pagamenti; anche questo va bene, ma già il decreto pone alcuni interrogativi: sono solo i Comuni che usufruiscono della sospensione dei pagamenti quelli che potranno godere degli aiuti alla ricostruzione? di predisporre una mappatura precisa dei Comuni che sono stati interessati dal terremoto del 24 agosto.

temporaneamente inagibili, con pochissimi interventi, anche non eccessivamente costosi, possono essere restituiti alle famiglie o, qualora pubblici, alla comunità.

di quantificazione del danno. Se il Governo o il commissario per il terremoto mi rivolgessero questa richiesta, potremmo dire - ad esempio - che nel mio Comune ci sono 2 milioni di euro di danni da sostenere. Potremmo già quantificare

le relative spese le copriremo in questa maniera. Ad oggi i Comuni interessati non dispongono neanche di un centesimo.